nuova finestra"). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Onorevoli colleghi e colleghe, comunico che il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato la seguente lettera: «Roma, 10 maggio 2016 Onorevole Presidente, informo la S. V. che il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data odierna, adottato su mia proposta, su mia proposta, ha nominato Ministro dello sviluppo economico il dott. Carlo CALENDA. F.*to* Matteo Renzi». Facciamo gli auguri di buon lavoro al nuovo Ministro. Informo che, come già comunicato ai Gruppi parlamentari per le vie brevi, nella seduta di *question time* di domani, alle ore 16, il ministro per gli affari regionali e le autonomie, onorevole Enrico Costa, risponderà a quesiti sui seguenti argomenti: stato del contenzioso sulla legislazione regionale; misure a sostegno della famiglia e della natalità.

codicistica e procedurale, relativamente alle procedure esecutive immobiliari. Quindi anticipo e comunico all'Aula questa intenzione del Movimento 5 Stelle e forse anche di altri Gruppi. lei sa che la Presidenza ha già preso posizione. Però credo che sia possibile che la Presidenza della Commissione giustizia chieda al Presidente del Senato di verificare ulteriormente. Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Anche noi, come Gruppo della Lega Nord, in Commissione abbiamo appena rilevato questa incongruenza, a nostro modo di vedere, sulla gestione dei lavori nella trattazione di questi importanti disegni di legge.

lo stesso processo di esecuzione forzata. Facciamo presente che, tra l'altro, il disegno di legge n. 2284, approvato dalla Camera dei deputati a marzo, che arriverà in Commissione giustizia, riguarda tutta la riforma del processo civile

che abbia un senso e un inquadramento all'interno del nostro ordinamento. Per questa ragione abbiamo fatto la richiesta in Commissione e auspichiamo che il Presidente della Commissione giustizia

e per ricordare a tutta l'Assemblea che stiamo parlando di un tema fortemente sensibile per tutta la popolazione. Stiamo parlando infatti di procedure esecutive e concorsuali

Grazie

Commissioni riunite. Abbiamo tremato di fronte alla possibilità che le esecuzioni immobiliari potessero diventare un fatto privato e gestito in esclusiva dalle banche. Ora non vogliamo certamente immaginare che il sistema della giustizia debba cedere in termini di garanzie, di certezza, di trasparenza per tutti gli operatori della giustizia, dagli avvocati a

misure a sostegno delle imprese e l'accelerazione del recupero del credito. Non vorremmo che il sistema della giustizia non fosse poi sufficientemente tutelante per tutti.

Signora Presidente, ho chiesto di intervenire per sottolineare un punto specifico del provvedimento al nostro esame, cioè l'inserimento,

per tutti i ragazzi che compissero nel 2016 i diciotto anni di età, anche ai ragazzi diciottenni, residenti in Italia, ma di origine non comunitaria. Nella finanziaria 2016 avevamo approvato una misura che riguardava non solo gli studenti italiani, ma anche gli studenti della comunità europea, ma avevamo impropriamente lasciato fuori questa fascia, anche numericamente contenuta, di ragazzi che spesso vivono nel nostro Paese,

Grazie ma che rappresenta, anche simbolicamente (ma non solo simbolicamente, perché 500 euro in tasca a un diciottenne possono rappresentare anche la differenza tra il potere andare a teatro oppure no, tra il poter acquistare un libro oppure no) un elemento di autonomizzazione dei ragazzi. Io da insegnante ricordo lo stupore dei miei alunni, quando li portavo in scambio culturale, magari in Paesi del Nord Europa come la Danimarca e la Svezia, e alle volte si trovavano a dovere condividere l'esperienza del dormire

Nel nostro Paese abbiamo poche misure che garantiscano ai nostri ragazzi una vita autonoma. Preferiamo mantenere l'idea che, all'interno della famiglia d'origine, si svolga un pezzo di *welfare* - e naturalmente va dato atto e va riconosciuto il valore di questo servizio che svolgono le famiglie d'origine - ma spesso si tratta di meccanismi che non agevolano l'autonomizzazione dei percorsi di vita dei giovani nel nostro Paese. Se vogliamo che i nostri giovani non vengano impropriamente accusati di eccessivo mammismo dobbiamo anche fare in modo che costruiscano la loro autonomia. Credo che questa possibilità di iniziare ad avere due soldi virtuali in tasca per costruire un maggiore spessore culturale in questa prima fase del loro percorso di autonomizzazione sia un fatto positivo. Volevo aggiungere solamente un'ultima considerazione. Fra i subemendamenti presentati all'emendamento del Governo, ce ne era uno della Lega in cui si chiedeva di subordinare

delle finalità, che sono propriamente quelle di produrre un maggiore livello di conoscenza della lingua, della Costituzione, delle istituzioni, della vita sociale, di come funziona il mercato del lavoro piuttosto che il sistema sanitario nel nostro Paese. Ritengo pertanto che sarebbe improprio

ai libri, quindi alla cultura - che può rappresentare uno di quegli strumenti finalizzati all'integrazione degli stranieri nel nostro Paese, così come previsto dallo stesso decreto sull'accordo di integrazione,

uno strumento che lo Stato mette a disposizione di questi ragazzi per far sì che quella integrazione avvenga meglio. Nel momento in cui stiamo discutendo - e spero arriveremo presto a definirla - della possibilità di ottenimento della cittadinanza da parte dei ragazzi stranieri che vivono nel nostro Paese, credo che questo sia un piccolo passo che va in quella stessa importantissima direzione. *(Applausi per i laghi di Levico e Caldonazzo, che mi sembra una cosa importante. *(Applausi)*. Salutiamo anche le studentesse, gli studenti e gli insegnanti dell'Istituto secondario di primo grado «Enrico Fermi» di Lusia, in provincia di Rovigo. Anche a voi benvenuti al Senato

Signora Presidente, eccoci di nuovo a parlare di scuola, a meno di un anno dalla concitata approvazione della riforma sulla esame, apparentemente innocuo: pochi articoli per prorogare i servizi di pulizia delle scuole affidati a società esterne e l'istituzione di una nuova università. Si tratta di un ennesimo provvedimento tampone per provare a risolvere i nodi non affrontati dalla buona scuola, a partire dai servizi di pulizia, di manutenzione quotidiana. Parliamo delle esternalizzazioni di servizi, di lavoro precario e di LSU mai assunti: oltre 21.000 persone, il 50 per cento delle quali si trovano nelle Regioni del Sud, disoccupati o cassintegrati che il Governo Prodi nel 2001 decise di stabilizzare all'interno delle scuole per i lavori di pulizia, ma nel 2007 le opere di pulizia furono sottratte agli enti locali per esternalizzarle. Sono seguite gare a ribasso, anche del 30 e 50 per cento, che hanno portato le ditte a ridurre gli orari di lavoro e le retribuzioni. Gli effetti sono evidenti a tutti: scuole poco pulite, poco manutenute, mansioni inappropriate e pericolose per i lavoratori. Il progetto scuole belle sono risorse per piccoli lavori di manutenzione con l'obbligo di farli attraverso le ditte di appalto pulizie o con il personale ATA, unico modo per garantire posti di lavoro. Eppure, la scadenza al 31 marzo di scuole belle ha portato alla procedura di licenziamento di 8.000-9.000 esuberi. Siamo dinanzi, dunque, ad una vera emergenza sociale e con questa proroga, però, dobbiamo dirci che semplicemente si rinvia il problema. Proroga che, tuttavia, Cantone (al quale il Governo ha affidato il senso etico e la legalità del proprio operato) ha messo fortemente in dubbio per evidenti illegalità. urgente per noi procedere a un piano straordinario di assunzione degli ATA, con la stabilizzazione di tutti i precari e la reinternalizzazione dei servizi di pulizia, perché dovete avere l'onestà di ammettere che le esternalizzazioni hanno fallito: hanno prodotto precarietà, aumento della spesa, peggioramento della qualità dei servizi e spesso corruzione. La presentazione del decreto-legge è stata tuttavia un'arma di distrazione per nascondere gli emendamenti della relatrice e del Governo che cercano di riparare ai danni e agli effetti della legge 13 luglio 2015, n. non è possibile reintrodurre le regole *ante* legge 107 senza sapere che, nel frattempo, gli effetti di quel provvedimento hanno avuto il loro esito. Il famoso comma 108 ha messo in moto un sistema e il solo fatto di cercare di cambiarlo

la discussione della riforma sulla buona scuola, ma eravamo stati tranquillizzati. Cosa è accaduto in questo anno scolastico è chiaro a tutti: sacrifici, tante malattie, aspettative, mille espedienti per poter giustamente ritornare a casa, ai propri figli e alla propria famiglia. una follia aver permesso tutto questo e figuriamoci se non è giusto dar loro la possibilità di riavvicinarsi a casa. Ma a quale prezzo e sulla pelle di chi? Ci sono circa 45.000 insegnanti delle GAE che non hanno fatto domanda di assunzione per non subire la deportazione nazionale. Cosa accadrà ora a tutti loro? Continueranno a lavorare con incarichi annuali o perderanno il posto? Verrà data loro la possibilità di fare domanda ed essere assunti perché nel frattempo sono cambiate le regole di ingaggio? *Divide et impera*. Questo esercizio arrogante del potere attraverso le assunzioni discrezionali è vergognoso. Abbiamo più volte denunciato che con la legge 107 non veniva fatta alcuna assunzione dei precari delle scuole dell'infanzia nelle GAE e che presto si sarebbe aperto un problema di giustizia sociale e carenza di personale nelle scuole. Il concorso è appena iniziato e a settembre non avremo i risultati per poter fare le assunzioni. Si accoglie allora un emendamento per le assunzioni di coloro che sono nelle graduatorie di merito 2012: un loro diritto, senza dubbio, peccato che si parli solo di Campania, Lazio e Sicilia. La magia delle elezioni fa dimenticare l'esistenza delle GAE. Avete la responsabilità di tenere ben aperta la guerra tra i precari perché vi siete rifiutati di fare un piano pluriennale per stabilizzarli. Ma voi preferite le questue, così potete concedere o meno il diritto al lavoro. Non abbiamo notizia sulla delega del progetto 0-6, ma un emendamento sostituisce la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi educativi con la definizione «bisogni educativi *standard*» perché - ci è stato detto - è l'Europa a chiedercelo. Vorremmo sommessamente ricordare che il tema dei livelli essenziali è richiamato dalla nostra Costituzione, in particolare dopo la riforma del Titolo V, per individuare unità, indivisibilità e fruizione egualitaria. Lo Stato individua i livelli essenziali per armonizzare il principio di autonomia e quello di uguaglianza, con un forte collegamento tra la prima e la seconda parte della Costituzione. Lo dunque, stabilisce le esigenze unitarie, valide per tutto il territorio nazionale, cui le Regioni devono attenersi nel momento in cui legiferano. Nel rispetto di quelle esigenze si può parlare, ad esempio, di scuole dell'infanzia e di asili nido. Si elimina, invece, il riferimento alla Costituzione e si introduce la definizione di bisogni educativi *standard*. Cosa sono? I bisogni *standard* sono gli indicatori economici che dovrebbero valorizzare efficienza ed efficacia dei costi, obiettivo di servizio cui devono tendere le amministrazioni locali definizione diversa dai livelli essenziali e allora crescono molti dubbi. State forse pensando di trasformare la fascia 0-6 in un servizio alla persona, piuttosto che un servizio a domanda collettiva? Parliamo di bisogni educativi *standard* per trovare, ad esempio, una copertura legislativa alla vergognosa operazione in atto a Firenze con l'appalto delle scuole dell'infanzia comunali ai privati? privati? Grazie ai continui tagli, anche vostri, lo Stato non è in grado di farsi carico delle scuole dell'infanzia comunali e così il Comune di Firenze sceglie di passare la loro gestione alle cooperative, sostituendo la figura dell'insegnante con quella dell'educatore. Ecco perché parliamo di bisogni educativi *standard*, altro che Europa. E magari pensate di elevare tutto questo a modello nazionale. Si sa che le risorse aggiuntive per questo Governo Governo si trovano, ma solo per le scuole private. Uno degli ultimi emendamenti presentati dal Governo ha previsto un ulteriore finanziamento alle scuole private per il 2017, in nome della presenza degli alunni disabili. È un tema serissimo che non può essere trattato con superficialità, intanto ricordare che lo Stato ogni anno versa alle scuole private 200 milioni, ai quali si sono aggiunti con la legge di stabilità 2016 altri 25 milioni; ben 225 milioni che sono già distribuiti con il criterio anche della disabilità. Di cosa parliamo allora? Nessuno è contrario agli interventi a sostegno della disabilità, ma qui è in discussione il drenaggio di risorse dalla scuola statale verso quella privata. Il fondo utilizzato è quello per le scuole statali, dove invece mancano gli insegnanti di sostegno per garantire il diritto allo studio costituzionalmente garantito ai ragazzi disabili. Non esiste alcun principio di uguaglianza nemmeno tra le scuole private. Le scuole private possono assumere da sempre gli insegnanti, anche di sostegno, e sarebbe grave se non lo avessero fatto in questi anni. Le scuole degli enti locali, invece,

Forse sarebbe utile destinare allora risorse alle scuole degli enti locali con questa finalità ben precisa e destinare ulteriori risorse all'assunzione degli insegnanti di sostegno per la scuola statale.

per molte settimane, non per l'ostruzionismo delle opposizioni, ma per i continui rinvii del Governo, che ha modificato continuamente il testo originale,

Nonostante tutto il tempo, nessuno spazio è stato lasciato a un confronto con le opposizioni; uno spazio vero per affrontare problemi reali. Tutte le volte che si parla di scuola troviamo conferma che l'ideologia dell'uomo solo al comando è preponderante e la democrazia diventa un orpello fastidioso, come dimostra l'ennesima fiducia che il Senato si accinge a votare, come stamattina ci ha preannunciato il presidente Napolitano. Signora Presidente, onorevoli colleghi, riservandomi di analizzare in maniera completa ed approfondita il decreto-legge in esame in sede dichiarazione di voto, voglio affrontare in questa intervento il tema specifico della scuola dell'infanzia e, in particolare, delle scuole paritarie.

è evidente e nota a tutti la grave difficoltà in cui versano per la situazione di bilancio tali scuole e la drammatica situazione che vede molte di queste costrette a cessare l'attività per l'impossibilità di chiudere i bilanci. Segnalo anche il caso del Veneto, sul quale richiamo l'attenzione proprio per la gravità che riveste: la dirigente regionale la settimana scorsa non ha avuto la garanzia di poter avere la dotazione organica necessaria per aumentare il numero di sezioni della scuola dell'infanzia statale per far fronte alla necessità di accogliere bambini che frequentavano scuole paritarie che hanno chiuso o che chiuderanno perché più nessuno è in grado di garantire il pareggio di bilancio. Se devo essere più esplicito, informo che dal prossimo anno scolastico, se persistesse l'attuale situazione, in alcuni Comuni ci sarebbero bambini che non potrebbero frequentare nel luogo di residenza la scuola dell'infanzia, a meno che i genitori non ricorrano a scuole pubbliche o paritarie di altri Comuni - non si tratta solo di Comuni minori - con evidente disagio e con maggiori oneri a carico delle famiglie. In tale contesto è apprezzabile, quindi, la previsione introdotta con un emendamento del Governo di assegnare un contributo alle scuole paritarie che accolgono bambini con disabilità. Nella situazione attuale queste scuole non hanno la capacità finanziaria per poter assumere insegnanti con le professionalità specifica per l'*handicap*, insegnanti che nella scuola pubblica sono garantiti dallo Stato, creando una evidente e ingiustificata discriminazione. Molte scuole paritarie sono, infatti, costrette a rifiutare l'iscrizione di bambini disabili. Questo quadro emerge dall'analisi dei dati sulle frequenze. Nella scuola pubblica il numero di alunni con disabilità è doppio rispetto a quello della scuola paritaria, e non si tratta di situazioni locali, in quanto è un dato che si presenta con la stessa caratteristica nelle varie regioni. Quanto proposto con il decreto-legge in esame è un primo, piccolo intervento a favore delle paritarie. È un punto di partenza e non può essere assolutamente la soluzione definitiva del problema. Con i 1.000 euro che sarà possibile erogare con l'istituzione del fondo di 12,2 milioni è impensabile, infatti, poter assumere un insegnante per tutta la durata di un anno scolastico. Anche la detraibilità della spesa nei limiti di 400 euro per ciascun figlio è stato un passo in avanti, troppo piccolo però per garantire la effettiva libertà di scelta dei genitori, prevista dalla Costituzione, nella frequenza scolastica dei figli. Non dobbiamo dimenticare che la legge n. 62 del 2000 ha creato i presupposti normativi per arrivare alla effettiva parità. Sono passati da allora sedici e poco, troppo poco, è stato fatto. Certamente non è colpa di questo Governo. La responsabilità ricade su tutti i Governi che dal 2000 si sono succeduti. A questo Governo che ha inteso intraprendere una strada nuova, che apprezzo, chiedo che nell'esercizio della delega affidata dalla legge n. 107, relativa alla scuola dell'infanzia, sia affrontata in maniera strutturale e definitiva la questione del sistema duale della scuola italiana in particolare, dell'infanzia. Non posso non richiamare che il costo che lo Stato sostiene per ciascun bambino che frequenta la scuola dell'infanzia pubblica è più che doppio rispetto a quello sostenuto dalla scuola paritaria. ricordo anche che il contributo che il MIUR assegna per ciascun frequentante è di 500 euro, mentre il costo per un bambino alla scuola pubblica è di poco inferiore a 6.000 euro annui.

deve far riflettere sulla inderogabile necessità di maggiore sostegno alle scuole paritarie. Per altre questioni contenute in questo decreto-legge mi riservo di intervenire in sede di dichiarazione di voto.

non sia presente in questa fase nella persona del Sottosegretario alla pubblica istruzione. Mi fido, però, del senatore Pizzetti che è attento alla discussione. Parlo dell'emendamento 2.201, che si sarebbe dovuto discutere in Aula e che riguarda l'articolazione del Fondo per il finanziamento ordinario dell'università, che raccoglie tutti gli atenei d'Italia sulla base di base di criteri definiti dal Ministero e che dovrebbero essere giusti. Voglio dire - tanto si parla molto di giustizia in quest'Aula - che la giustizia non è solo quella che si fa nei tribunali. La giustizia è anche quella che si fa con gli atti di Governo e che si fa in questo Parlamento: è giustizia nel senso più alto del termine, cioè quella che rende giusta una società, che non discrimina.

e, sulla base della definizione di popolazione studentesca, si assegnano gli stanziamenti a ciascuno degli atenei. Per l'Italia centrale la popolazione studentesca vale 30 milioni di abitanti, per l'Italia insulare, la nostra, vale molto ma molto meno, perché siamo 1.600.000 abitanti. Le università nella penisola sono avvantaggiate nei criteri e, quindi, prendono più soldi. scippando una quota di finanziamenti agli atenei sardi sulla base di questo criterio, perché

E siccome è considerato un punteggio aggiuntivo avere Regioni contermini, essendo la Sardegna un'isola, di contermine ha il Mar Mediterraneo che - com'è noto - non ospita popolazione, neppure studentesca. Il risultato di questa vicenda è che 4, 5, 6 milioni di euro nel 2016 saranno scippati alla Sardegna e dati alle altre università nazionali. E questo lo sa benissimo il Ministero, visto che ha incontrato i rettori di Sassari e Cagliari e il Presidente della Regione; ha assunto un impegno e ha fatto questo provvedimento, ma quell'impegno se l'è già rimangiato, perché non c'è una riga sull'argomento. Adesso voi farete il maxiemendamento, farete il maxiemendamento, nel quale ripristinate il finanziamento almeno del 2015 per il 2016 per la Regione sarda; fatelo con questo contenuto perché dentro quel fondo i soldi ci sono e non possono essere prelevati sempre da una

Strano, tutto questo è molto strano, anche perché, a quanto pare, al Governo della democrazia e del lavoro di Commissione non interessa, e ciò è grave.

Tutto questo è assurdo. Ad ogni modo, il testo ha due termini: proroga e stabilizzazione. La proroga è per il programma delle scuole belle, ma chiunque va a vedere che cosa sono le scuole, le nostre scuole, si accorge che di bello non hanno niente, a partire dalla soglia per entrare al loro interno, così come i giardini, i muri, le vetrate, gli infissi, i soffitti e i controsoffitti. Io che ho avuto la possibilità di girare le classi, ho visto le aulette dei bidelli dove c'erano i bidoni delle vernici e gli stucchi pronti per essere utilizzati per stuccare il soffitto,

di sostegno. I 12 milioni vengono, quindi, aggiunti agli ulteriori 500 milioni annui alle scuole paritarie, togliendo valore al fondo che serve per le scuole pubbliche, il Fondo per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione. Tutto questo non serve al futuro del nostro Paese e non fa altro che far crollare il nostro Paese nella realtà. Qui si parla di cose belle, di cose belle, di scuola buona; si parla nella finzione, perché nella realtà è tutto molto diverso.

colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, con la conversione in legge del decreto-legge n. 42 del 2016, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca, troviamo affrontato un tema, all'articolo l, relativo a urgenti disposizioni per il decoro degli edifici scolastici e per lo svolgimento di pulizia e servizi ausiliari nelle scuole. Durante questa discussione

una situazione che non va relegata a *slogan* e a deleterie semplificazioni per rispetto soprattutto delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti. In coerenza con il piano straordinario sull'edilizia scolastica, in due anni sono stati avviati oltre 12.000 interventi - come si può vedere sul sito, e i dati sono forniti dalla cabina di regia - suddivisi in scuole nuove, scuole sicure, scuole innovative e scuole belle. Il e scuole belle. Il decreto-legge si riferisce in particolare al ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, rispetto al quale si è raggiunto un accordo, siglato l'8 marzo 2016, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le organizzazioni sindacali e i rappresentanti dei consorzi aggiudicatari degli appalti Consip; accordo in cui il Governo si è impegnato a sostenere la prosecuzione del programma sino alla data del 30 novembre 2016, mediante lo stanziamento di ulteriori 64 milioni di euro nell'anno 2016.

sono, quindi, evidenti nel primo articolo, così come appaiono manifesti rispetto al secondo articolo, quello relativo alle disposizioni per la stabilizzazione e il riconoscimento della scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute.

Certo, questo tema ha anche aperto una discussione più generale sulle politiche della ricerca, in merito alla quale la 7a Commissione del Senato si è spesso confrontata, ipotizzando forme di coordinamento utili a sinergie e valorizzazione della qualità. I passaggi emendativi hanno arricchito questo decreto-legge di ulteriori contenuti che si riferiscono a situazioni contingenti di altrettanta rilevanza. Per brevità ne cito alcuni che ritengo meritori di sottolineatura, ben sapendo che molta attenzione si è riversata sulle misure urgenti in materia di assegnazioni provvisorie del personale docente in ruolo. La *ratio* - come è stato detto - è tendere alla maggiore prossimità rispetto ai territori di residenza dei docenti, nel momento in cui sceglieranno definitivamente la cattedra. Così come molta attenzione - e si rivelerà una misura efficace - è giusto porre sulle disposizioni riguardanti i docenti della scuola dell'infanzia, prevedono che i docenti inseriti nelle graduatorie di merito del 2012, non assunti nei ruoli regionali per incapienza, possano essere assunti in Regioni diverse da quella per cui hanno concorso nel limite massimo della percentuale non superiore al 15 rispetto ai posti disponibili per ciascuna Regione. Un decreto ministeriale di emanazione del MIUR entro trenta giorni dalla conversione del presente decreto-legge definirà i termini e le modalità riferibili anche all'ordine di preferenza tra tutte le Regioni del sistema scolastico statale che i docenti dovranno indicare. Particolarmente degno di nota è il dispositivo riguardante gli incarichi di supplenza breve o saltuaria, sui quali sappiamo si sono verificati gravi ritardi di pagamento degli stipendi. Tale aspetto

ogni opportuna forma di cooperazione al fine di garantire, ciascuna per la propria competenza, la tempestiva assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche e il pagamento mensile delle somme spettanti al personale a tempo determinato per le prestazioni di lavoro rese. Il Consiglio dei ministri, di concerto con il MIUR, adotta entro sessanta giorni apposito decreto per la definizione dei termini specifici. Il pagamento deve comunque avvenire entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno del mese di riferimento. Al fine di meglio gestire tale problema, al personale supplente docente o ATA è assegnato un codice identificativo identificativo univoco, che accompagna la vita del supplente fino - si spera - all'immissione in ruolo che tutti si auspicano, al fine di ottimizzare e semplificare le procedure di gestione di stato giuridico del personale scolastico. Nel decreto-legge è contenuto anche l'incremento di 8 milioni di euro per i compensi

in ragione della condizione di disabilità nel calcolo dell'ISEE, anche ai fini del riconoscimento di prestazioni scolastiche agevolate. È una misura, questa, di massima urgenza e fortemente attesa dai portatori di interesse, nonché da tanti studenti che vedono riconosciuto il diritto allo studio.

definisce i destinatari della carta elettronica del valore di 500 euro in un modo diverso. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale a tutti i residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità,

carta può essere utilizzata per assistere a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'acquisto di libri, nonché per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e spettacoli dal vivo. Le somme assegnate con la carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario, a proposito del discorso relativo all'ISEE. Proprio lunedì, a Roma, l'associazione Save the Children, in occasione della campagna «Illuminiamo il Futuro» ha presentato il rapporto «Liberare i bambini dalla povertà educativa: a che punto siamo?». È un tema che abbiamo affrontato anche nel nel quarto piano nazionale per l'infanzia e nella legge di stabilità con disposizioni anche importanti sul piano dell'allocazione di risorse.

Questo provvedimento conferma ancora una volta l'attenzione del Governo, e sicuramente di quest'Aula, alla qualità della scuola di cui la nostra società ha estrema necessità; una scuola che, nel processo di acculturazione e formazione per tutti, vede la chiave per costruire un presente e un futuro basato sulla cittadinanza attiva, consapevole della propria identità e per questo dialogante, democratica e inclusiva.

Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato con grande attenzione il dibattito e anche gli autorevoli contributi che sono stati offerti dalla senatrice Cattaneo e dal presidente emerito Napolitano, in particolare sui temi della ricerca. Personalmente condivido molti dei temi posti sulla necessità di rilanciare innanzi tutto la ricerca,

abbiamo scritto anche, come Partito Democratico e come forze della maggioranza, diversi documenti e proposte che credo il Governo stia valutando. Non so se il termine «agenzia» in questo Paese a volte faccia venire i brividi alla schiena,

Abbiamo chiari quali siano i problemi: pochi laureati rispetto agli obiettivi di Europa 20-20, un insufficiente collegamento con il mondo del lavoro, mobilità sociale stagnante, forte contrazione del personale docente e insufficiente numero di ricercatori

tra scuola e università; insufficienza di alternative di formazione terziaria non universitaria. Dopo i 3 miliardi all'anno investiti nella legge di stabilità del 2015 con la buona scuola e con la legge di stabilità 2016, sono arrivati

È stato avviato il piano straordinario di 6 milioni di euro (poi 10 milioni per il 2017) per l'assunzione di professori di prima fascia. Ci sono 25 milioni di euro per la quota premiale delle università

sono stati lo sblocco totale del *turnover* per i ricercatori più giovani, quelli di tipo A, e il consolidamento per sempre, con un investimento di 86 milioni di euro nel 2013, di 6.000 contratti per gli specializzandi di medicina, che ridurranno la forbice tra immatricolati Fra le cose fatte c'è anche la riattivazione, dopo tempo, del bando PRIN 2015, con 92 milioni per la ricerca di base del sistema pubblico. Sono già arrivate oltre 4.000 proposte, la cui valutazione si chiuderà in autunno. Quanto al progetto Human Technopole Italia 2040, varato con il decreto-legge n. 185 del 2015, sappiamo che sono attese a giorni le osservazioni sul progetto da parte del *panel* di esperti internazionali indipendenti, a cui si è rivolto il Ministero si è rivolto il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per avere una valutazione imparziale e qualificata sul progetto di realizzazione di un polo tecnico‑scientifico nell'area Expo 2015. Il comitato scientifico è guidato dall'Istituto tecnologico di Genova, che voglio ricordarlo - è sì una fondazione di diritto privato, ma i cui soci sono pubblici e, dunque, perseguono finalità di tipo pubblico. tecnologico ha redatto il progetto, accoglierà le osservazioni del comitato internazionale e consegnerà il *masterplan* definitivo a Palazzo Chigi; dopodiché, nei provvedimenti che seguiranno, questo Parlamento sarà pienamente coinvolto. Come si sa e come avete ricordato, esso prevede un investimento decennale di circa un miliardo e mezzo e il reclutamento di 1.500 ricercatori, 1.000 di *staff*, tra i quali 150 ricercatori *technology* e 400 PhD,

CNR. Il grande polo scientifico tecnologico milanese si focalizzerà sulla comprensione della correlazione fra nutrizione genomica, invecchiamento e aspettativa di vita, nella direzione di quella che viene definita «la medicina di precisione». L'obiettivo generale è, infatti, quello di utilizzare la genomica, i *big e le nuove tecniche di diagnostica per sviluppare approcci personalizzati, per affrontare in particolare i tumori e le malattie neurodegenerative, per mettere capo a nuovi approcci di biotecnologia applicati anche all'agricoltura. Sono tutti temi su cui ci sono una vocazione e eccellenze nel nostro Paese. In questo progetto sono, quindi, coinvolte fondazioni e aziende, per attrarre investimenti privati e fungere il prima possibile da incubatore di *start up*.

I sette centri in cui si articolerà saranno supportati da tre servizi di facilitazione, utilizzati da tutti gli scienziati del Technopole*:* il primo riguarderà una piattaforma di genomica, il secondo un centro di *imaging* e il terzo un ambizioso centro di *data storage and high performance computing*.

particolare ai quesiti della senatrice Cattaneo, se pensiamo che la ricerca sia un elemento essenziale per la crescita del Paese, occorre una visione di sviluppo verso cui tendere

i Governi possono giocare un ruolo importante nel sostenere la nascita di un *cluster*, che poi ovviamente devono continuare a sostenere. Certo, servono politiche, leggi e regimi fiscali favorevoli, adeguate politiche anche sui permessi di soggiorno per coloro che accogliamo nel nostro Paese Il successo di un progetto di ricerca non dipende solo da quanto si investe, ma anche dalle persone e dalle persone e dalle relazioni che riescono ad instaurare. Ecco perché si è scelta un'area in cui concentrare un investimento e un *network* ampio di ricercatori e di relazioni tra ricercatori e industria. Servirà certamente

Voglio poi rispondere ad alcune sollecitazioni o forse a delle provocazioni contenute in altri interventi, come quello del senatore Centinaio. Devo dire che il suo sembrava più un intervento rivolto al proprio Governo. I tempi della carta igienica da portare a scuola sono finiti. Gli 8 miliardi di euro li avete tagliati voi: qui si sono investiti 3 miliardi all'anno e 126 milioni di euro

Signor Presidente, onorevoli colleghi, innanzitutto vorrei ringraziare qui oggi la relatrice e tutti i componenti della Commissione per il lavoro che è stato svolto su questo disegno di legge. Anche il dibattito in Aula è stato costruttivo, importante e contribuisce sicuramente al lavoro del Governo che ritiene l'istruzione e la ricerca fondamentali per il Paese. Come già evidenziato da molti colleghi, il decreto-legge interviene su alcuni punti fondamentali, quali la proroga del programma scuole belle e - come è già stato detto in quest'Aula è importante perché garantisce la funzionalità delle scuole. Vi è poi la stabilizzazione dell'Istituto Gran Sasso, Grazie

Il decreto-legge interviene anche su altri argomenti: si prevedono - ad esempio - misure urgenti per gli alunni con disabilità. Come ha evidenziato il senatore Conte, in molte Regioni le scuole paritarie offrono il 66 del servizio e, quindi, è importante garantire a esse la possibilità di accogliere i bambini disabili. Come sapete, l'intervento è minimale: si garantiscono mille euro circa per bambino. I bambini disabili delle scuole paritarie oggi sono circa 12.000.

la possibilità di accedere alla cultura e a tutto quanto contribuisca a farli migliorare e integrare nel Paese civile che li ospita. Si modifica l'attuale disciplina in materia di ISEE per garantire e escludere dal reddito disponibile, oggetto della dichiarazione, i trattamenti economici percepiti dai soggetti con disabilità in ragione della loro condizione. Nell'ambito della discussione generale, questa mattina, alcuni colleghi hanno sollevato questioni relative al progetto Human Tecnopole. Desidero sottolineare innanzitutto come il Governo abbia inteso raccogliere la grande eredità di Expo, che ha portato a Milano studiosi di tutto il mondo a confrontarsi sui temi dell'alimentazione e dello sviluppo sostenibile. Tali concetti trovano un momento di sintesi nella Carta di Milano. Il Governo ha, quindi, previsto un primo stanziamento di 80 milioni per raccogliere proprio quanto Expo ha prodotto, e che non deve essere dimenticato, al fine di costituire a Milano un polo di ricerca internazionale. In tale quadro, è stato chiesto ad IIT di svolgere un ruolo di capofila, in considerazione del profilo di eccellenza

che i sette direttori dei centri di ricerca saranno selezionati sulla base di bandi internazionali da subito, secondo procedure *standard* di *call* internazionale. Contestualmente, si provvederà a costruire un *board* di indirizzo che consentirà di garantire una *governance* istituzionale, rispetto alla quale la partecipazione del MIUR assicurerà il raccordo con il sistema universitario e della ricerca italiano. Con riferimento alla valutazione del progetto, evidenzio come sono stati individuati nove valutatori, tutti operanti all'estero, dagli Stati Uniti, al Giappone, passando per la Germania e il Regno Unito. Il criterio utilizzato per individuare i valutatori è

Una volta ricevuti tutti i riscontri da parte dei valutatori internazionali, IIT provvederà a rivedere il progetto, per tenere conto dei commenti-suggerimenti e arrivare così ad un progetto definitivo da sottoporre al Governo. Ci aspettiamo che questo processo possa essere concluso entro poche settimane. Il progetto completo, a quel punto, sarà reso pubblico, e saranno resi pubblici anche i giudizi dei valutatori: ognuno potrà, quindi, farsi un'idea di come i giudizi degli eminenti scienziati internazionali, alla guida di alcuni dei centri di ricerca più prestigiosi al mondo, siano stati integrati nella versione finale del progetto. È già previsto, quindi, che tutto ciò avvenga nella massima trasparenza, secondo quanto è prassi nella comunità scientifica internazionale a cui il progetto si ispira dal primo giorno della sua ideazione. Il Governo è naturalmente disponibile a fornire, ove richiesto nelle opportune sedi parlamentari, tutte le informazioni che saranno ritenute necessarie.

è reduce dall'aver fatto l'identica cosa alla Camera dei deputati, ponendo la fiducia su un provvedimento che non è stato possibile votare in Senato neanche una volta. Si è potuto votare la fiducia e basta: non un voto in Commissione, non un voto in Sulla scuola si è potuto fare qualcosa di più, però ci risiamo: siamo ancora in una situazione in cui non si possono approfondire i problemi. Strano che poi le leggi non funzionino! Oggi affrontiamo il problema delle scuole. Quest'anno le scuole avranno forse la carta igienica, ma chi parla con il il personale, le famiglie e gli studenti sa che le scuole versano in una situazione di grave carenza. Eppure si sono trovati i soldi per finanziare con 60.000 euro ogni posto di lavoro guadagnato con il *jobs act*,

impegna il Governo a rispondere alle interrogazioni su cui ha un arretrato clamoroso, di gran lunga peggiore di quello di tutti i Governi precedenti. Non abbiamo nessuna traccia.

e sta creando, soprattutto sul sistema scolastico, sconcerto e disorientamento, tutti aspetti molto lontani dalla patina del tutto pubblicistica di efficacia, prontezza e soluzione dei problemi. Sulla scuola non c'è stata soluzione di problemi. Sulla scuola è piombata una cappa di disinteresse generale e gli insegnanti sostanzialmente sono stati lasciati soli. Oggi, con la richiesta di questa fiducia, li si schiaffeggia una volta di più, perché una volta ancora li si lascia soli e si impedisce a parlamentari eletti e legittimamente chiamati a rappresentare la volontà dei cittadini che li hanno eletti

l'educazione, di tacere e di non chiedere alla scuola di continuare a dare, quando non le si dà neanche la dignità di essere rappresentata con un percorso parlamentare serio.

assistiamo, in questa ultima fase, a una degenerazione nella proliferazione dei voti di fiducia. Questo non Questo non può essere addebitato esclusivamente a questo Governo, perché è una prassi che nelle ultime legislature ha subito degli aumenti esponenziali progressivi, con tutti i Governi, con i Governi di centro-sinistra e centro-destra. Cambiava la tipologia di Governo; venivano disattesi il più delle volte anche i richiami dell'alta magistratura dello Stato. Ricordo, ad esempio, le precise puntualizzazioni del presidente Napolitano quando faceva riferimento a un'altra prassi assai preoccupante: il treno della decretazione d'urgenza usato per

esimere dal cercare di mettere un attimo di attenzione sulla materia in esame. Il fatto che le cose siano andate in questa maniera, in coincidenza con una riforma costituzionale che obbliga tutti noi a un maggiore tasso di virtù per il futuro, ci impone, a mio parere, di riflettere sulla necessità di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

una nuova finestra"). La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione dei lavori sulla questione di fiducia posta dal Governo sull'emendamento interamente sostitutivo del disegno di legge di conversione del decreto-legge sulla funzionalità del sistema scolastico e della ricerca,

sugli effetti finanziari del maxiemendamento, il tempo è stato ripartito in un'ora e quindici minuti in base a specifiche richieste dei Gruppi. Le dichiarazioni di voto avranno luogo domani mattina a partire dalle ore 9,30 e a seguire ci sarà la chiama, orientativamente intorno alle ore 11. a seguire ci sarà la chiama,

l'emendamento 1.900 e ha riscontrato che esso riproduce integralmente il testo approvato dalla 7a Commissione,

ha riscontrato anche che la relazione tecnica, regolarmente bollinata da parte della Ragioneria generale dello Stato, esprime parere di nulla osta senza alcuna condizione.

Signor Presidente, colleghe e colleghi, signori del Governo, la richiesta di non passaggio agli articoli è stata motivata con argomentazioni puntuali e precise, anche con il senso profondo di uno sdegno, che si è avvertito negli interventi dei colleghi e in particolare del collega Malan, che ha ricordato come ormai vi sia una marginalizzazione progressiva dell'attività del Parlamento, che vede sempre di più ridursi il perimetro entro il quale svolgere le proprie prerogative, che sono anche legislative. Pare però che il Parlamento sia ormai definitivamente commissariato dal Governo, non soltanto sul versante della funzione legislativa, Grazie dall'inizio del Governo presieduto da Matteo Renzi - ma anche nella sempre più evidente compressione compressione tra il ricorso alla decretazione d'urgenza, più volte sottolineato come metodo abusato da parte del Governo, e il conseguente voto di fiducia, che evidentemente

di idee e di valutazioni, talvolta aspre, ma molto spesso orientate all'individuazione della strada più vicina ad intercettare il bisogno della gente.

colleghe e colleghi - e ci dispiace moltissimo - neanche quando è di tutta evidenzia che non c'è un atteggiamento pregiudizialmente negativo nei riguardi del Governo. Il fascicoletto degli emendamenti presentati al provvedimento in questione, che snocciola - per così dire - un lavoro ridotto all'osso e che si riassume in meno di cento emendamenti, non ci racconta di un atteggiamento ostruzionistico delle forze politiche di opposizione; tutt'altro. In quegli emendamenti si rintraccia la laboriosità del Parlamento, il desidero e la voglia di partecipare per correggere e portare un contributo al miglioramento dei testi. Poi dobbiamo fare i conti con la sconsolante valutazione che ci viene dal giudice amministrativo prevalentemente quando si trova a dover valutare l'inadeguatezza

un prodotto legislativo che faccia chiarezza e vada nella direzione di risolvere i problemi del Paese. sarebbe veramente auspicabile un'inversione di tendenza. Ho sentito l'intervento del collega Casini, il quale ha fatto appello a un atteggiamento di maggior equilibrio da parte del Governo. E noi avremmo accolto volentieri un atto di resipiscenza *in articulo mortis*, perché sarebbe stato veramente lodevole da parte del Governo emendare se stesso ed evitare che la politica del presto e male ancora una volta in quest'Aula accompagnasse, come il feretro verso l'ultimo viaggio, verso il viale dei cipressi, alla consegna di un prodotto che naturalmente è destinato soltanto a creare la rovina e lo scempio di un Paese che è allo stremo. Concludo, perché è anche utile uscire fuori Grazie dalla Commissione con tanto di disco verde del Governo, recante per titolo «scuole di specializzazioni non mediche», è il più grave insulto che viene fatto dal Governo e dall'Aula, se, con il voto fiducia, approverà questo scempio, perché sostanzialmente tradisce se stesso. Mi fa piacere che in Aula ci sia il sottosegretario D'Onghia che per competenza sovrintende a queste problematiche. l'articolo 2-*bis*, che viene introdotto con l'emendamento che ho citato, fa riferimento alla possibilità di una deroga alle norme sulla definizione delle scuole di specializzazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riferendosi

in modo assolutamente errato - mi permetto di dire volutamente errato e spiegherò il perché - sono invece disciplinate dal recente decreto interministeriale n. 68 del 4 febbraio 2015, su cui è accaduto il miracolo, perché si è creata una proficua sinergia e convergenza di vedute tra il Ministero della salute, il MIUR e il MIUR e il Ministero dell'economia. Qual è il motivo per il quale si fa questa truffa ai danni dei professionisti? Perché li si vuole sottrarre dall'obbligo che il Governo ha - e che costoro fanno bene a reclamare come diritto - di riconoscergli la borsa di studio: parliamo delle professioni di odontoiatria, di farmacista e di fisico medico. medico. Questa è la modalità con cui il Governo opera. Io dico che bisognerebbe incominciare a provare il senso della vergogna quando ci si presenta con provvedimenti di questo genere, li si approva con il voto di fiducia, espropriando il Parlamento del proprio ruolo e soprattutto non consentendo al Parlamento di poter proporre, in modo intelligente, proficuo, propositivo e utile per la comunità, degli elementi correttivi. Siccome è evidente che il Governo vuole andare avanti da solo e non vuole assolutamente che si disturbi il manovratore, a noi non resta che esprimere il nostro deploro

"scuole belle", ovverosia quella serie di norme che, nelle intenzioni del Governo e del Ministero della pubblica istruzione, dovranno rendere le scuole agibili, sicure e meglio conformate alle esigenze didattiche. debba continuare a essere finanziato anche per i prossimi anni credo sia cosa giusta e opportuna, ma, se ci è consentito, dobbiamo muovere due rilievi. Il primo è relativo ai 20.000 operatori, lavoratori socialmente utili, che, nell'ambito di questo provvedimento, sono già stati utilizzati all'interno della scuola

perché in questa scuola qualcuno cominci a pensare anche a queste figure di supporto, e non solo a implementare la platea dei docenti. Lo diciamo anche perché ci siamo fatti dei conti. L'accordo che il Governo ha stipulato l'8 marzo 2016 con le organizzazioni sindacali prevede che di questi 20.000 lavoratori socialmente utili

L'importo a carico della previdenza sociale per dare la cassa integrazione a queste persone per il biennio 2014-2016 ammonta a circa 45 milioni di euro;

invece di caricare sull'erario 45 milioni di euro di debito, in un bilancio di 850 miliardi di euro non si riescano a trovare appena altri 21 milioni

deve farsi carico delle spese sostenute, non venendo rimborsato neanche di un centesimo. Tutta questa storia

che credo costeranno svariate decine di miliardi di euro, si dovrebbero trovare anche qualche centinaia di milioni

Grazie

Grazie

Se gli elementi positivi complessivamente prevalgono, non si può, comunque, tacere il fatto di trovarsi di nuovo di fronte all'ennesima ripetizione del dilemma del parlamentare che, Grazie Può cadere un Governo per la scuola sperimentale di dottorato del Gran Sasso? Ovviamente no. Ci sono responsabilità enormi di fronte a una questione di fiducia che spostano l'attenzione dal merito del provvedimento alle alle implicazioni istituzionali che un voto negativo avrebbe. È chiaro che, di fronte a questa responsabilità, bisogna pensare al Paese nel suo complesso. Però è frustrante che non ci sia la possibilità di una discussione ed è frustrante, ogni tanto, la protervia con cui le scelte vengono giustificate. È veramente difficile, quando si vuole cercare di spostare qualche piccolo elemento all'interno di un provvedimento, confrontarsi con questa tecnica legislativa. Non dico niente di nuovo; lo sappiamo tutti in questa Aula, ma che il problema ci sia e che prescinda dal colore delle maggioranze politiche non può essere taciuto. Far finta che sia tutto bello e che funzioni tutto bene mi sembra un'ipocrisia alla quale non mi voglio associare. Nel merito, dicevo prima, prevalgono gli elementi positivi. Sicuramente è condivisibile l'obiettivo generale del provvedimento, che è quello di sostenere e migliorare il funzionamento complessivo del sistema scolastico e di ricerca. Sappiamo tutti che ce n'é un bisogno disperato; basta vedere il dato dell'OCSE rispetto al numero dei laureati e dei dottori di ricerca in Italia per rendersene conto. È molto importante, positivo e fondamentale il fatto che ci sia una sorta di partita di giro e uno sblocco rispetto al patto di stabilità, ma in ogni caso sono dei soldi che vengono mossi e messi in circolazione.

sia per quanto riguarda la maggiore chiarezza dei requisiti per l'attività di supplenza, sia per l'introduzione e il perfezionamento dei sistemi di valutazione dei dirigenti scolastici, la previsione di una loro responsabilità e di criteri meritocratici e la previsione di corsi professionalizzanti per alcune categorie professionali come agrotecnici, geometri, periti agrari e industriali, rispettando e, forse, incremento l'autonomia della singola università per quanto riguarda la concessione dei crediti formativi.

quando si mettono in circolazione dei soldi per la cultura va bene a prescindere dalle eventuali intenzioni nascoste dei proponenti. Questa è sempre una cosa positiva. Il punto critico principale nel merito riguarda in generale la politica della ricerca che non

non è accettabile che siano reperite risorse, in questo caso per la stabilizzazione e il riconoscimento di una scuola sperimentale di dottorato internazionale, riducendo le risorse disponibili dai fondi ordinari,

di un'iniziativa complessiva per la ricerca scientifica e tecnologica cui far partecipare tutte le università e i centri di ricerca, pubblici, privati e quant'altro? È una decisione che non mostra una grande logica alla base rispetto a una coerenza del sistema della ricerca complessivo. In terzo luogo, come ha detto il presidente Napolitano, non vi sono state delle sedi di confronto su questa materia. le risorse pubbliche in un settore strategico come quello della ricerca sono poche, devono essere per l'appunto soggette a una riflessione maggiore di quella che, pur rispettandone i contenuti, viene fatta all'interno dei Ministeri. L'altro profilo problematico riguarda i contributi alle scuole paritarie. Qui sappiamo che, rispetto all'articolo 33 della Costituzione, ci sono delle letture storicamente contrastanti. La mia lettura può essere diversa rispetto a quella che si è imposta nella dottrina e poi nella prassi politica maggioritaria. Resta nel complesso positivo l'intento di sostenere gli alunni con disabilità anche nelle scuole paritarie. In ogni caso, l'obiettivo è positivo. che ha suscitato polemiche il criterio di ridefinizione dell'ISEE per i nuclei familiari che abbiano persone con disabilità, tanto più perché non ha tenuto conto di un recente intervento del Consiglio di Stato. L'auspicio è che, dovendo comunque mettere mano di nuovo, in modo complessivo, a una riforma del sistema di detrazione e di franchigie lo si possa fare tenendo maggiormente in conto tutte le varie voci degli interessati, che sicuramente possono avere molto da dire anche per esperienza diretta. Quindi, per concludere, poiché prevalgono complessivamente gli aspetti positivi nel merito, pur con tutti i mal di pancia che derivano da un modo di procedere che sicuramente non è particolarmente gratificante per il ruolo di noi tutti all'interno di quest'Aula, e siccome il voto di fiducia va letto comunque alla luce delle conseguenze che questo potrebbe avere, è chiaro ed evidente che il senso di responsabilità, oltre che la condivisione sostanziale di larghe parti del provvedimento porterà ad esprimere un voto favorevole. PRESIDENTE.

Io vorrei intervenire su ciò che c'è in questo decreto-legge, ma anche su ciò che non c'è, signor Presidente. Vorrei farlo anche alla luce dell'apposizione della fiducia sul maxiemendamento interamente sostitutivo, proprio perché alcune questioni, che io ritengo fondamentali specialmente nel campo della ricerca, proprio a causa della questione di fiducia sono state soppresse. Erano presenti, ad esempio, degli emendamenti che affrontavano alcune questioni specifiche, su cui tornerò a breve.

una nuova università per decreto-legge, invece di avviare grandi dibattiti e grandi discussioni su cosa sia meglio fare e sia meglio creare. Inoltre, come è stato già sottolineato, il finanziamento stesso di questa nuova università, esaminando la copertura stabilita dal Governo, incide sul finanziamento ordinario degli enti di ricerca. Sostanzialmente la torta è sempre la stessa e si fanno delle fettine sempre più piccole, erodendo il monte complessivo dei finanziamenti al settore della ricerca. Quindi, già intravediamo pertanto alcune problematiche significative rispetto a questo *modus operandi*. Tali problematiche sono notevolmente accentuate dal fatto che vi erano degli emendamenti,

rendeva il merito una caratteristica predominante nell'attribuzione delle risorse. Si è deciso che quel modello non funziona più, perché l'università e gli enti pubblici di ricerca sono dei carrozzini pubblici soggetti a tanti vincoli, che non funzionano e i cui finanziamenti si reputa non siano efficaci. efficaci. Sostanzialmente si vuole passare a un nuovo modello di politica della ricerca, che vede entrare in campo dei nuovi soggetti, di natura privata e di diritto privato, perché il privato viene visto come sinonimo di efficienza, quindi un modello aziendalistico anche nella ricerca,

prevedeva un finanziamento decennale fino al 2014, che però è stato prorogato. Oggi ci troviamo in una situazione in cui soltanto l'1 per cento del bilancio di quell'ente (bilancio tra l'altro neanche pubblico, quindi per

pubblici di ricerca, con un piano assunzionale altamente insufficiente di 1.000 ricercatori e di 500 "cattedre Natta", la cui somma ammontava a circa 95 milioni di euro. Ebbene, noi stiamo dando a questa fondazione di diritto privato, che è già piena di soldi, quasi lo stesso ammontare che abbiamo dato a tutte le università e a tutti gli enti pubblici di ricerca. Pertanto, signor Presidente, quando dico che stiamo spostando il fuoco della politica della ricerca in Italia, lo dico con cognizione di causa,

questa percentuale sarà destinata ad aumentare se non fermiamo immediatamente questa deriva, questo modo di fare politica della ricerca in Italia. Ebbene, a fronte di tali osservazioni, la replica della relatrice Puglisi e del sottosegretario

Quindi, sostanzialmente questi soci pubblici non li vedo. Si tratta di un consiglio direttivo formato prevalentemente da soggetti privati, che gestisce dei soldi pubblici in modo totalmente oscuro, non rendicontato, con una giacenza tra l'altro estremamente grande. Inoltre, la Commissione bilancio - e mi rivolgo anche al presidente

che timidamente (ma è di gran significato) si è lamentato dell'ennesima fiducia e del fatto che un ordine del giorno di cui si faceva latore (quasi come i capitolari carolingi *ad personam*, non certo strumenti democratici di un Paese occidentale e democratico come il nostro) non venisse accolto dal Governo perché purtroppo c'era l'ennesima fiducia. Sono seguiti altri interventi, che protestavano e si lamentavano di questo; ha protestato il senatore Casini, sempre in modo mite, per carità, per non turbare troppo

tutto, anche sulle riforme che avrebbero avuto bisogno principalmente di una discussione in queste Aule, di un confronto tra parlamentari, che sono, poi,

Fuori da quest'Aula tutti voi, colleghi, siete d'accordo nel dire che mai come in questa legislatura si è avuta una decretazione così sproporzionata; ma non è una piccola aberrazione del sistema: è la fine di un sistema democratico. Non è colpa del Governo, ma del Parlamento, perché non esistono i padroni se gli schiavi non vogliono. senatrice Mussini)*. Non è solo l'ennesima, velata polemica sul malfunzionamento di questa democrazia: voi avete permesso che si mettessero i ceppi e il guinzaglio alla democrazia parlamentare e che oggi si conduca al patibolo questa democrazia. Non è solo questione di riforme: qui si tratta di riforme costituzionali di iniziativa del Governo e di leggi elettorali su cui avete messo la fiducia, di temi etici come le unioni civili su cui avete messo la fiducia. Non è soltanto l'arroganza del Governo:

Quindi perché non far votare questo Parlamento? C'è qualcosa che va oltre il Signor Presidente, gentili colleghi, con questo intervento desidero esprimere la piena solidarietà, come Gruppo Italia dei Valori, al procuratore capo di Napoli, Giovanni Colangelo. È infatti notizia di questi giorni, come saprete, la rivelazione di un pentito della sacra corona unita, che ha portato alla luce un piano organizzato dalla camorra per attentare alla vita del procuratore. Sono stati anche sequestrati, giorni fa, 550 grammi di tritolo, che dovevano servire a questo scopo, prova quanto mai inquietante dell'attendibilità delle rivelazioni del pentito. Siamo di fronte a un fatto di una gravità inaudita volto a colpire un servitore dello Stato, che in questi anni combatte, insieme ai suoi colleghi, per estirpare la camorra e contrastare la criminalità da un territorio che vive la speranza di un diverso futuro. Un uomo che, oltre al coraggio e al senso del dovere, ha dimostrato in questi anni di saper condurre una strategia efficace e che ha idee precise su come migliorare ancora la lotta contro la criminalità organizzata sia quella che spara al rione Sanità (per usare le sue parole) sia quella che punta agli appalti e che si infiltra nelle istituzioni. Non dobbiamo quindi abbassare il livello di attenzione e sottovalutare queste minacce. Ancora oggi il terrorismo più pericoloso nel nostro Paese è quello delle mafie e dei corrotti.

Signor Presidente, vorrei riprendere una cosa che ho sentito questo pomeriggio dal collega Malan il quale, attingendo ad una notizia comparsa ieri a caratteri cubitali su «Libero», ha fatto riferimento a 100.000 posti di lavoro fasulli che sarebbero stati prodotti della riforma del lavoro che abbiamo varato lo scorso anno. «Libero» fa riferimento, stravolgendoli, ai dati forniti dall'INPS, che non parlava affatto di posti di lavoro fasulli ma, al contrario, di

100.000 nei quali l'INPS ha contestato all'impresa la regolarità della fruizione della decontribuzione stessa. Quindi i posti di lavoro esistono eccome e sono basati su contratti a tempo indeterminato, producono reddito e gettito contributivo e non sono in nessun modo qualificabili come posti di lavoro fasulli. Colgo l'occasione per osservare che ogni giorno che il buon Dio manda in terra i giornalisti, giustamente, rimproverano a noi politici

Grazie